Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti

4.0.202 (già 4.0.5), 7.0.200 (già 7.0.23), 8.204 (già 8.66), 9.0.2, 14.0.1, 18.211 (già 18.8), 24.0.200 (già 24.0.2), 24.0.4, 28.0.3, 30.0.6, 32.0.200 (già 32.0.4), 33.201 (già 33.12), 33.0.201 (già 33.0.3), 34.0.200 (già 34.0.2), 38.0.200 (già 38.0.5),

(già 47.0.8), 48.0.200 (già 48.0.1), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5. La Presidenza dichiara altresì improponibile l'emendamento 39.0.200 e inammissibile

nel merito vorrei far presente che la maggioranza ha accolto un mio ordine del giorno, poi accolto come raccomandazione, in relazione ai crediti di carbonio e all'impronta di carbonio. È molto importante mettere in relazione questi due aspetti affinché siano monitorati con attenzione, perché è un meccanismo che va a compensazione. Invito il Governo ad accogliere anche quest'ordine del giorno in merito ai crediti di carbonio e all'impronta di carbonio.

51.200 è di natura *bipartisan* e fa riferimento al cosiddetto Repower EU, e cioè alla parte supplementare che comunque segue le regole del PNRR, ieri più volte citato dal Ministro. Con tale emendamento chiediamo che i circa 5 miliardi di spesa che possono essere aggiunti sotto forma di Repower EU siano oggetto di relazione e di approvazione da parte del Parlamento entro giugno. Ci sembra che questa iniziativa serva a rimettere in pista i fondi aggiuntivi Repower EU esattamente con le stesse prerogative e gli stessi obblighi che hanno riguardato tutte le quote relative al PNRR. Sarebbe strano che una quota, per quanto piccola, ma significativa, del PNRR che si aggiunge, ossia circa 6 miliardi, fosse sottratta sia all'obbligo di trasparenza che naturalmente c'è in tutte le parti che riguardano il PNRR, sia alla prerogativa del Parlamento di potersi esprimere e approvare. Credo che questo sia un punto che riguarda tutto il Parlamento e tutte le forze politiche. Mi meraviglierei se il Governo e anche i colleghi della maggioranza volessero esprimersi contro questa richiesta di trasparenza, responsabilizzazione del Governo e prerogative del Parlamento.

è l'aumento dell'occupazione femminile e giovanile. Non è un obiettivo scontato e lo abbiamo ottenuto grazie a una mobilitazione e a impegni che quest'Assemblea anche nella scorsa legislatura, in modo unitario, ha preso sull'occupazione femminile come grande obiettivo del Paese. dell'Unione europea siamo il Paese con il tasso di occupazione femminile più basso. I dati dell'Istituto europeo per la parità di genere relativi al 2022 ci posizionano al quattordicesimo posto e sull'occupazione siamo tra i peggiori.

Il decreto-legge n. 77 del 2021, all'articolo 47, prevedeva delle linee guida per l'applicazione di tale clausola. Le analisi ci dicono che troppe stazioni appaltanti stanno andando in deroga a quella clausola che prevede il 30 per cento di occupazione femminile e giovanile nel PNRR. Chiediamo quindi una relazione sugli effetti e sull'applicazione della clausola di condizionalità e sull'impatto di genere *ex ante* ed *ex post* dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Io credo che non possa essere una richiesta solo dell'opposizione: è un obiettivo del Paese, oggi davanti a noi, che fa innalzare il PIL della nostra Nazione e non solo. L'occupazione femminile è un veicolo di sviluppo per tutti, anche per gli uomini, e comporta ricchezza. È chiaro che non si ottiene solo con la clausola. È per tale ragione che abbiamo voluto il Fondo per le infrastrutture sociali e i servizi educativi zero-sei; tutte misure che noi continuiamo a chiedere come obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

stazioni appaltanti e delle imprese sull'applicazione della clausola di condizionalità per l'occupazione femminile e giovanile. Sottolineo che tale emendamento è in funzione anche della discussione che abbiamo svolto ieri sulla questione della coesione sociale:

dell'energia, impegna il Governo a valutare nel capitolo REPowerEU, integrativo del PNRR, di prevedere specifici stanziamenti destinati al finanziamento di strumenti di incentivazione di tipo fiscale che, al pari di quelli previsti dalle misure Industria 4.0 e formazione 4.0 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 23, siano in grado di promuovere ulteriormente gli investimenti finalizzati alla realizzazione di processi produttivi verdi, sostenibili e resilienti.

il Governo a valutare nel capitolo RepowerEU, integrativo del PNRR, di prevedere

«impegna il Governo: a garantire la continuità operativa delle amministrazioni centrali titolate al monitoraggio del PNRR e all'attuazione di specifici investimenti e riforme; adoperarsi per garantire la piena attuazione, nel rispetto degli obiettivi europei e nazionali, tanto del PNRR quanto del PNC, con particolare riferimento ai profili finanziari, tenendo conto dell'aumento del peso dei *target* rispetto alle *milestone* previsto per i prossimi mesi; a garantire una maggiore accessibilità ai dati relativi all'attuazione del PNRR, con particolare riferimento alle piattaforme a ciò preposte, a iniziare da "Italia domani"; a garantire il pieno raggiungimento delle priorità trasversali connesse al Mezzogiorno, ai giovani e alle donne».

«impegna il Governo a monitorare affinché vengano concretamente attuate le previsioni del nuovo codice degli appalti relative alla riduzione della garanzia fideiussoria alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere e all'impegno per tutti gli operatori economici, nella fase di esecuzione del rapporto, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione sociale per le persone con disabilità o svantaggiate, nonché alla possibilità, per le stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, il raggiungimento dei predetti obiettivi, con particolare riguardo agli appalti la cui partecipazione o esecuzione è riservata a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle predette persone». G1.203, con la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza, i trasferimenti alle Regioni destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10

a spendere in modo efficace i soldi del PNRR sia ripristinare Impresa 4.0, rafforzandola con un grande piano ambientale e di risparmio energetico, con l'incentivazione cioè di tutti i beni che ricadono in queste categorie. Ciò prevede una spesa rapida, effettuata dalle imprese, in modo che tali soldi non si perdano. Su questo chiediamo al Governo di esprimersi. Riteniamo che ciò derivi dal modo in cui a nostro avviso si deve fare opposizione, e cioè proponendo sempre e non solo protestando, perché questo è il senso del lavoro che facciamo in questa sede. Questa è la nostra proposta, di cui abbiamo parlato col Governo. L'abbiamo presentata

dati aggiornati rispetto a quelli che invece sono stati poi esplicitati dalla Corte dei conti. Speriamo che con quest'ordine del giorno il Governo provveda a far sì che tutti i dati siano resi disponibili, come prevede la legge, in maniera tale che vi sia un controllo sociale esterno e non soltanto di queste Crediamo che si possa anche inserire il punto che garantisce il recupero degli obiettivi su giovani e donne. In ogni caso, con la richiesta che venga ripreso anche quest'ultimo punto, accogliamo la riformulazione

parere è contrario. L'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, al fine di favorire l'applicazione - in condizioni di certezza operativa - delle discipline previste dal piano Transizione 4.0, stabilisce che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione.

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge n. 132 del 2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Sì, Presidente, insisto e chiedo anche di conoscere possibilmente la motivazione del parere contrario. Stiamo parlando di dotare gli enti di ricerca e le università di personale per supportare il raggiungimento degli obiettivi legati al PNRR e al PNC. Pertanto, non si capisce come mai questa maggioranza dica a parole di volere

maggiori risorse per il personale degli enti di ricerca e delle università per le finalità legate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del PNC. Nell'attesa di sapere se il Governo ci vuole ripensare,

che anche gli altri enti di ricerca che ricevono un finanziamento diretto dai Ministeri, come quelli che hanno un finanziamento diretto dal MUR, possano beneficiare di tutto quell'*iter* semplificativo per la rendicontazione. chiedendo semplicemente che non ci siano oneri dal punto di vista fiscale e dal punto di vista finanziario per gli enti di ricerca pubblici che hanno finanziamenti dai Ministeri. Chiediamo di sapere il motivo di questa distinzione fra gli enti di ricerca che sono controllati dal MUR e gli enti di ricerca che hanno finanziamenti da altri Ministeri.

nel rispetto dei vincoli di bilancio, un piano triennale di assunzioni a valere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 diretto a consentire l'assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 così come modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

vorrei sottolineare come in Commissione abbiamo preso atto del parere contrario del Governo su un emendamento che amplia le semplificazioni anche ai piani regionali integrati energia e clima (PRIEC), che sono gli unici piani che al momento ci sono. Pertanto, se tutto quel pacchetto di semplificazioni non è attuato anche sui PRIEC è come se non ci fosse quindi, con alcuni colleghi delle forze politiche di maggioranza, ci sembrava che ci fosse un possibile ripensamento del parere su questo emendamento, su cui noi voteremo a favore. Chiedo però una riflessione anche alla maggioranza, perché significa ampliare le semplificazioni previste anche ad altri piani credo che ciò vada nell'ottica di accelerare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non capiamo oggettivamente le ragioni del parere contrario.

stipulati finora per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee verrebbero modificati e si creerebbe un contenzioso tra le imprese e i proprietari dei terreni. Se viene modificata la normativa sulle aree idonee, infatti, capite che in questa fase transitoria si potrebbe creare un problema. Quindi, l'emendamento 47.230 fa sì che in una fase transitoria le aree idonee, fino a nuova normativa, rimangano quelle stabilite dalla precedente norma. Non capisco perché sia stato espresso un parere contrario, quando l'emendamento è di buon senso.

preciso e puntuale, le norme sugli impianti fotovoltaici, anche considerato il fatto che le aree idonee ancora non sono perfettamente definite a livello nazionale. Vedo quindi una

Governo,

«Il Senato, premesso che appare necessario garantire il coinvolgimento del Parlamento in merito all'aggiornamento del PNRR e all'utilizzo dei nuovi fondi del capitolo Repower EU, previsti per accelerare la transizione energetica, impegna il Governo: a predisporre e a inviare al Parlamento una relazione illustrativa degli investimenti e delle riforme inserite nella proposta di aggiornamento del PNRR che include anche quelli relativi al capitolo Repower EU».

Signor Presidente, che gioia in questo macello! Facciamo un attimo scemare il disastro?

Signor Presidente, Ministri, colleghi senatori e senatrici, la terza rata del PNRR ci sarà, anche se in ritardo. Non è un'eccezione, lo abbiamo fatto anche con altri Paesi. Quello che è cruciale è la dimensione del programma a sostegno della ripresa italiana. È così importante che un impegno congiunto di Bruxelles a Roma dovrebbe essere fondamentale, se si vuole attuare questo Piano. A pronunciare queste parole è stato non il *premier* Giorgia Meloni o il ministro delegato Fitto o qualche sospetto segretario politico di maggioranza, ma il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, espressione non a caso del PD,

tutte le inutili e improduttive polemiche sollevate dall'opposizione negli ultimi giorni e ieri in quest'Aula, nonostante peraltro una rara sincerità della politica, quella del ministro Fitto, che ha denunciato le difficoltà oggettive di realizzare tutte le opere previste dal PNRR per i mali atavici del nostro Paese. Vorrei sapere chi dei colleghi dell'opposizione può smentire, Presidente, la dichiarazione secondo cui l'intero ammontare delle risorse del PNRR non potrà avere completa attuazione entro il 2026, se non si apportano alcune modifiche al Piano, con la Commissione europea che ci è venuta incontro con il RepowerEU e che ci dice che c'è l'esigenza di modificare il PNRR. Avendo un Governo che, piaccia o meno, ha davanti l'orizzonte di una legislatura, è responsabile voler capire subito se ci sono progetti che non potranno essere realizzati entro il 2026. Invece di fare squadra in Europa, l'opposizione cosa fa? Parla di contrapposizione tra MEF e Presidenza, perché il Governo ha fatto la scelta di mettere in campo un Ministero per l'attuazione del PNRR, riscontrando l'esigenza ovvia di un luogo di coordinamento e di assunzione di piena responsabilità nell'attuazione di un programma da 220 miliardi di euro, per evitare le modalità precedenti che hanno portato alla realizzazione di soltanto circa il 34 per cento dei progetti. Il MEF mantiene - ci mancherebbe - tutta la parte del monitoraggio e dell'attuazione della parte finanziaria del programma, propedeutica all'inoltro delle richieste di rata di finanziamento alla Commissione europea. Vorrei che fosse chiaro dunque agli italiani che ci ascoltano, con questa premessa, che oggi stiamo convertendo non semplicemente il terzo decreto-legge in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per farci capire dagli italiani, ai quali questo acronimo è ostico, si tratta di 220 miliardi per l'Italia che tutti sogneremmo, un nuovo rinascimento italiano, il futuro nostro e dei nostri figli, la nostra fama internazionale di capacità di fare del bello, la dignità di Paese fondatore dell'Unione europea e membro del G7 e del G20; un'Italia all'altezza e locomotiva dell'Europa, moderna, ricca di infrastrutture produttive, digitale, sostenibile, cablata, riforestata, all'avanguardia, *green*, efficace ed efficiente, come dice il ministro Fitto. Da quello che ho sentito in quest'Aula, non credo che le opposizioni lo abbiano capito o, peggio, che a loro interessi capirlo, anziché fare solo polemica - in un momento nel quale è necessario invece fare squadra ed essere, opposizione e maggioranza, la nazionale ideale del nostro Paese.

Chiarisco anche, a scanso di equivoci, che concordiamo col Governo che non si debba perdere neppure un euro rispetto a quelli assegnati, ma che per farlo dobbiamo coinvolgere il privato, dando i soldi agli italiani, non come con il reddito di cittadinanza, per essere chiari, con un fondo che è presente in ogni Paese del mondo, un prestito d'onore agli italiani, che implica non lacci e lacciuoli burocratici, ma la verifica che i fondi vengano spesi in maniera corretta, a pena di galera. Una volta certificata l'impossibilità di rubare, siamo certi che gli italiani saranno capaci di moltiplicare i soldi, per le capacità creative che che abbiamo e che sono riconosciute nel mondo. Almeno 20, di quei 220 miliardi di euro, dovrebbero essere dedicati agli italiani e la Commissione europea non potrà dire di no, visto che la finalità del PNNR, per chi non lo sapesse, è creare ricchezza. Ovviamente, non parliamo di aprire un bar, ma di progetti di carattere innovativo. Faccio un esempio: se un privato assume la responsabilità di interrare con una sua azienda tutta l'alta tensione nazionale, fa un investimento di bellezza, già fatto in Francia, avendo noi tutti i nostri punti più belli del Paese devastati dai tralicci. Questo è nell'interesse del Paese e della bellezza, quindi si tramuta in un volano per l'economia e il turismo italiani. Il decreto-legge contiene misure molto importanti, che vanno da una nuova *governance* ad altre misure di notevole portata, che riguardano la pubblica amministrazione, la scuola, i commissari del Governo che potranno sostituirsi eventualmente agli enti locali in caso di inerzia o di ritardi, ai provvedimenti di semplificazione delle procedure, al dimezzamento delle tempistiche per gli appalti e così via.

Governo Meloni - che io chiamo codice Frattini e che ricordo è stato scritto non da Meloni o Salvini, ma da un *pool* di giudici espressione della più alta magistratura, coordinato appunto dal compianto presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini. Troviamo scorretto anche colpevolizzare il precedente Governo guidato da Mario Draghi, il quale si trovò un piano già redatto dal Governo giallorosso di Conte. Draghi ha avuto appena un mese di tempo per correggere gli errori tecnici, le manchevolezze e le inadeguatezze tecniche e giuridiche presenti in quel testo che, se non corretti, probabilmente ci avrebbero condotti condotti dritti a una clamorosa bocciatura da parte della Commissione. Certamente, trenta giorni di tempo sono stati un lasso troppo esiguo per porre mano anche ai progetti relativi a un'infinità di piccole opere sparse su tutto il territorio nazionale, affidate perlopiù a piccoli enti locali sprovvisti di personale di personale adeguato per attuarle. Allo stesso tempo, per rispetto della verità, è corretto affermare che le problematiche che si riscontrano sul PNNR sono state ereditate dal Governo Meloni e che non sono assolutamente figlie di scelte di questo Esecutivo: non dirlo sarebbe negare l'evidenza. Il Piano - non bisogna dimenticarlo dimenticarlo mai - fu scritto in un contesto storico completamente diverso dall'attuale. Non si può non tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'inflazione, dovuti essenzialmente al Covid e soprattutto al conflitto in Ucraina, che hanno giocato un ruolo a dir poco perverso soprattutto nel settore dei lavori pubblici. Ancora, non si può non chiedere un attento riesame di talune opere, che oggettivamente appaiono superate o non rispondono più alle esigenze attuali, né alla prospettiva di centrare l'obiettivo della transizione ecologica, energetica e tecnologica del Paese, cui l'intero PNNR è finalizzato. In questo senso, crediamo fortemente nell'idea manifestata dal ministro Fitto di tenere in conto per l'Italia non solo i 191 miliardi di euro del PNNR, ma anche i 30 del Piano complementare, che sono risorse nazionali, e gli 80 miliardi di euro delle risorse UE, relative al periodo 2014-2020, non spese. Si tratta complessivamente di oltre 300 miliardi di euro. Crediamo infine sia passata inosservata o sia stata poco considerata l'idea manifestata dal Presidente della Corte dei conti europea, Tony Murphy, in un'intervista a «Il Sole 24 Ore» Ore» che, dopo aver notato le evidenti difficoltà delle amministrazioni locali italiane, alle prese con la gestione di una massa di denaro mai giunta in queste dimensioni, ritiene che le istituzioni europee potrebbero prendere in seria considerazione l'ipotesi di concedere più tempo all'Italia per la realizzazione del PNNR. Per l'autorevolezza di chi l'ha presentata, questa idea non va fatta cadere, signor Ministro. In conclusione, noi siamo molto fiduciosi che, nel negoziato con l'Unione europea, si troverà il modo di fronteggiare le difficoltà e di modificare il Piano.

quasi che il Governo non rappresentasse l'intero Paese. Invece, sarebbe utile avere un dialogo serio, con il Governo e la maggioranza, fondato sulla concretezza, senza pregiudizi e strumentalizzazioni. È in gioco il futuro dell'Italia e degli italiani. L'argomento è fin troppo importante per interpretarlo in modo sbagliato. In ogni caso, la maggioranza, di cui il Gruppo che ho l'onore di rappresentare è parte, andrà avanti, con coraggio e determinazione, avendo come stella polare l'interesse esclusivo e generale dei cittadini, in particolare dei nostri giovani e dei nostri figli. Il Governo, anche in questa circostanza, può contare sul nostro convinto sostegno. *(Applausi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, vorrei iniziare questo mio intervento cercando di precisare che, per quanto riguarda il lavoro in Commissione, anche da parte mia vi è stato il riconoscimento di una grande correttezza da parte del presidente Calandrini. Vorrei dire al ministro Fitto che, per quanto ci riguarda, abbiamo però coerentemente votato contro e che

volevano affrontare e hanno affrontato temi quali la *governance*, sulla quale lei ci ha spiegato ieri che quello che è stato fatto e che avete deciso è stato concordato con Stato e Regioni.

ma a me non pare che ci stiamo andando. Ad esempio, il Mezzogiorno è sparito dall'agenda politica. Eppure, è la grande questione che non da oggi, ma da sempre il nostro Paese

lavoro è una spesa, ma ha una resa, perché ha un futuro dal punto di vista della costruzione della nostra società e dello sviluppo. Come si fa, ad esempio, nella pubblica amministrazione, a trattenere i tecnici che hanno una certa professionalità? Intanto, rinnovando i contratti. Sottolineo che nel settore sanitario i contratti sono fermi: è stato rinnovato quello del 2019 fino al 2021, ma siamo nel 2023 e non si parla

sta avvenendo un fatto grave nella sanità, ovvero che molti operatori medici e paramedici se ne vanno e diventano contrattualisti.

sviluppo economico. È una discussione che abbiamo fatto anche sul superbonus e poi sui crediti incagliati; per cinque mesi siamo andati avanti, ma parliamoci chiaro: come si fa a rilanciare l'occupazione locale in questo Paese? Ad esempio, nel settore dell'edilizia, se interveniamo sul terreno della

e che vanno in una certa direzione. Si produrrebbero rigenerazione urbana, rivalorizzazione del proprio patrimonio e messa sul mercato di appartamenti a costi accessibili che possono essere anche elementi di calmierazione dei prezzi, con la possibilità per le nuove generazioni di staccarsi dalla famiglia e di fare molte cose. Ora però bisogna avere un'idea di Paese e capire che Paese vogliamo, perché a me pare

mi aspetto almeno che faccia la destra sociale e invece voi avete sposato un'impostazione prettamente liberista, che guarda molto alla grande impresa e ai grandi profitti; altro che dare risposta ai problemi sociali! Questa è la contestazione che noi rivolgiamo ed è per questo che come Alleanza Verdi e Sinistra voteremo convintamente contro il disegno

come Gruppo per le Autonomie abbiamo apprezzato il contributo del ministro Fitto in Commissione bilancio e anche alcune sue precisazioni in Aula nella replica di ieri pomeriggio, anche se rimane certamente qualche scollamento fra le dichiarazioni di principio e i contenuti normativi che ci apprestiamo ad approvare. In una sorta di eterogenesi dei fini, la dichiarata volontà di accelerare e semplificare l'attuazione del Piano può invece realisticamente tramutarsi nell'indebolimento della struttura di *governance,* nella sua perdita di efficacia e con essa nell'impossibilità di ottenere i primari obiettivi economici che il PNRR si prefiggeva: migliorare i livelli e i tassi di crescita del PIL e assicurare la sostenibilità del debito pubblico. Il PNRR, oltre ad essere un piano di investimenti da 191,5 miliardi, cui si sommano i 30 miliardi del Fondo complementare nazionale, oltre ad essere un Piano di riforme strutturali e uno straordinario progetto politico, dev'essere considerato come l'ultima grande occasione per modernizzare il Paese, persa la quale difficilmente l'Italia potrà recuperare il *gap* che la separa dagli altri Stati europei e occidentali. Mi riferisco ai *gap* relativi ai profili infrastrutturali, digitali, energetici e *green,* ma anche alla coesione sociale.

e, dall'altro, accentrandola nell'ispettorato generale per il PNRR presso il MEF, rende necessario che i passaggi di consegne avvengano il più rapidamente possibile, per evitare di perdere tempo prezioso. Altrimenti, intervenendo in questo modo, il Governo rischia concretamente di rallentare l'azione amministrativa proprio nel momento cruciale della messa a terra di investimenti e riforme. Questa sola prima argomentazione è di per sé sufficiente a indurci a definire questo decreto-legge come parzialmente inopportuno. Il secondo motivo di preoccupazione riguarda la trasformazione della corretta tensione alla semplificazione in una sorta di pericolosa *deregulation,* con il rischio di sottoporre a minori controlli la legalità, la salute, la sicurezza e l'impatto ambientale; ma non basta, perché le novità normative critiche riguardano anche l'eccesso di accentramento con un abuso del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi. Il terzo punto debole riguarda l'assenza di un forte affiancamento a favore degli enti locali, destinatari del 20 per cento dei fondi, pari a 40 miliardi per cento dei progetti e il 42 per cento del finanziamento delle misure ad oggi ripartite vedono come soggetto attuatore i Comuni. La quasi totalità degli enti comunali risulta coinvolta nelle iniziative del Piano. Tuttavia, resta incerta la capacità di spesa delle amministrazioni comunali, in particolare di quelle che negli anni hanno registrato bassi livelli di investimento per mancanza di risorse, ma anche per difficoltà gestionali, per carenza di personale e di competenze tecniche; un'incertezza che aumenta con riferimento ai territori del Mezzogiorno in cui maggiori sono i divari territoriali da colmare. nonostante il Dipartimento per le politiche di coesione attesti che il 41 per cento delle risorse sia stato formalmente assegnato al Mezzogiorno, permangono timori circa la capacità di completare la fase di attuazione degli interventi entro il 2026, in un contesto segnato da tempi di realizzazione delle opere pubbliche storicamente superiori a quelli medi nazionali. Non è certamente sufficiente prevedere premi di produttività per il raggiungimento degli obiettivi a dirigenti e segretari comunali, se primariamente non vengono rinforzate le strutture con personale avente adeguate competenze e formazione specifica. Infine, l'intenzione del Governo di una verifica a livello nazionale sulla fattibilità delle centinaia di interventi previsti e la trattativa con Bruxelles per la rimodulazione del Piano non rappresentano gli atteggiamenti responsabili di chi vuole evitare ritardi, ma anzi sono in se stessi ostacolo alla positiva conclusione del Piano. La proposta di rinunciare a una parte dei fondi a debito è evidentemente insostenibile per la maggioranza, proprio perché contiene in sé due evidenze: la prima, i 122 miliardi costituiscono non nuovo debito, ma in gran parte mera sostituzione del finanziamento di interventi già previsti - penso tra tutti alle misure 4.0 - con finanziamento più conveniente, perché garantito dalla tripla A europea. La seconda evidenza è che la rinuncia agli interventi del PNRR impedirebbe il raggiungimento dei livelli e dei tassi di crescita del PIL già previsti ed essenziali per i conti nazionali. Nessuno che abbia a cuore il futuro dell'Italia rallenterebbe e depotenzierebbe nei fatti la realizzazione del PNRR, a meno che il vero obiettivo del Governo non sia, in realtà, politico-elettorale e guardi dritto alla preparazione della propaganda per le europee del prossimo anno. Quale miglior obiettivo può infatti esserci che non quello di colpire direttamente il cuore della Next generation EU, proprio quel programma comune che ha permesso all'Europa, per la prima volta dalla sua costituzione, di ragionare e agire come un'unica entità politico-istituzionale che sceglie di assumere debito comune europeo e che scommette sul cammino verso l'unica modernità europea, fatta di medesime libertà e valori, di minori disuguaglianze, di maggiore coesione e di grandi transizioni strategiche? Aggiungo e con questo concludo - che, nonostante la massiccia propaganda fatta a favore dell'autonomia differenziata, questo Governo non ha nemmeno voluto accogliere l'emendamento delle autonomie speciali che chiedevano di fare ciò che è naturale: rispettare le competenze di programmazione delle autonomie e permettere che fossero non i singoli o i piccolissimi Comuni a doversi occupare direttamente dei bandi e della messa a terra del PNRR, bensì direttamente le Province autonome di Trento e Bolzano. L'intento e la dichiarazione tracciata dal presente decreto-legge non sono completamente condivisibili e sono potenzialmente pericolosi per l'Italia, per la sanità pubblica e per le autonomie locali.

Signor Presidente, colleghi, con il decreto-legge in esame il Governo interviene sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche sul Fondo complementare e sulle regole delle politiche di coesione. Lo fa assumendosi le proprie responsabilità, com'è giusto che sia. Da un lato, in modo condivisibile, prova a continuare con la strada che il Governo Draghi aveva già intrapreso, quella di una profonda semplificazione; dall'altro lato, si assume la responsabilità di rivedere complessivamente la *governance*. È un provvedimento ampio, di fronte al quale avremmo potuto scegliere una linea di opposizione dura, rimarcando contraddizioni, debolezze e incertezze che pure non sono mancate. Noi invece preferiamo uno stile e un'impronta diversa. Semplicemente, vi mettiamo in guardia su un rischio che intravediamo all'interno di questo provvedimento, ovvero che la scelta legittima del Governo di rivoluzionare la *governance*, consentendo a ciascun Ministero di ripensare le strutture di missione del PNRR in un anno cruciale per la messa a terra degli investimenti più importanti, possa determinare non un accelerazione del Piano, ma un suo rallentamento. Ci sono anche alcune scelte che fatichiamo a comprendere: innanzitutto, la scelta che avete fatto, per una ragione di consenso, di prendere tempo sui balneari, cercando di raccontare un rinvio *sine die* di gare che invece ci saranno e rispetto alle quali sarebbe più corretto, nei confronti di quelle imprese, dire la verità e fare in modo che quegli imprenditori e quelle famiglie comincino ad attrezzarsi rispetto a uno scenario ineluttabile. Dall'altro lato, ministro Fitto, mi lasci dire che impiegare tre Consigli dei ministri per varare il disegno di legge annuale per la concorrenza ci lascia un po' sbalorditi *(Applausi)*, perché la legge per la concorrenza è uno dei provvedimenti fondamentali del PNRR. Quindi, c'erano anche le argomentazioni per poter fare un'opposizione dura, ma noi abbiamo scelto un approccio diverso, perché il PNRR, anche nell'avvicendarsi dei Governi, per noi resta una straordinaria opportunità per l'Italia. Non è mai stato il piano Conte o il piano Draghi e per noi oggi non è il piano Meloni: è il piano dell'Italia e per l'Italia. È la speranza viva di poter finalmente modernizzare questo Paese, di superare i divari Nord-Sud e di rimettere al centro il tema della salute che, dopo la pandemia, sembra un po' offuscato, ma resta un problema gigantesco di liste d'attesa, di medici che non ci sono e di infermieri che mancano. *(Applausi)*. Sono 230 miliardi e per noi, Ministro, non sono troppi. Per una vita ci siamo lamentati dei tagli e dell'assenza delle risorse. Oggi abbiamo 230 miliardi e qualcuno nella sua maggioranza riesce a dire che sono troppi. Trovo che sia una polemica un po' fuori luogo, perché quei soldi rappresentano investimenti che dovrebbero portare non solo a una modernizzazione del Paese, ma anche a una nuova idea d'Europa. Non vanno sprecati e non saranno mai per la nostra visione oggetto di una strumentalizzazione politica. Per questo, Ministro - come ha fatto ieri la collega Fregolent - torno anch'io a un ringraziamento nei suoi confronti, perché abbiamo apprezzato la disponibilità all'ascolto all'ascolto e al confronto, che ha portato dei risultati. Meglio sarebbe stato secondo noi non stravolgere la *governance* del Piano, non ne ravvedevamo la necessità. Tuttavia, se volete farlo, fatelo. Delle scelte però che state compiendo vi dovete assumere la responsabilità fino in fondo. Quindi, non potete giocare allo scaricabarile, non ci sono più alibi, ma ci sono le scelte che avete assunto e che riguardano anche le politiche di coesione. Ministro, ha illustrato una relazione nella quale risulta che su 126 miliardi, 65 dei quali cofinanziati con i fondi strutturali europei, le risorse spese sono 43 miliardi. È un dato certamente non soddisfacente. La domanda che ci poniamo però è se, per invertire questa tendenza cronica, la strada giusta sia quella adottata dal Governo. La soppressione dell'Agenzia di coesione con il trasferimento delle funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione è una scelta forte, su cui attendiamo il Governo alla prova dei fatti e alla capacità di spesa integrale di queste risorse. Con riferimento ai ringraziamenti, dicevo prima che ci sono emendamenti frutto di un lavoro svolto dai colleghi Lombardo e Paita in Commissione bilancio e aggiungo che ci sono emendamenti importanti. Sicuramente un passo nella giusta direzione è stato compiuto rispetto a Italia Sicura,

È sicuramente un buon passo avanti. Viene poi parificato il regime giuridico dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato, favorendo un altro passaggio molto importante, quello verso la ricerca dell'impresa. Vi è un emendamento positivo per quanto riguarda le strutture residenziali universitarie e vi sono anche delle semplificazioni richieste per l'installazione di impianti fotovoltaici. Infine, c'è un ordine del giorno che impegna il Governo a rivedere, all'interno del Repower EU, la possibilità di utilizzare una parte delle risorse del PNRR per una misura di successo, Industria 4.0 *(Applausi)*, voluta dall'allora ministro Carlo Calenda e che, attraverso quest'ordine del giorno, vogliamo estendere all'ambito della transizione ecologica, della transizione digitale e della formazione. Resta il capitolo delle riforme, di cui si parla meno, ma che agli occhi della Commissione europea e soprattutto per il futuro dell'Italia non è meno importante. Presidente, che il tasso di riformismo di questo Governo è ancora tutto da dimostrare, perché, al netto delle parole e del tentativo di uscire dall'angolo inventando qualche nuovo reato ogni volta che c'è una difficoltà *(Applausi)*, ci sono provvedimenti che languono.

il *made in Italy* è un bello *slogan* che viene però portato avanti dalla capacità delle nostre imprese e non da un sostegno forte da parte delle istituzioni e del Governo. non dirsi liberali, ma essere nei fatti favorevoli alla concorrenza. *(Applausi)*. Su questo non c'è solo il nodo dei balneari, che meritano trasparenza rispetto alle criticità che le loro imprese devono affrontare, ma anche le gare per la distribuzione del gas, per i servizi pubblici locali *(Applausi)* e per gli ambulanti. Vi invito quindi a fare presto anche da questo punto di vista. Vi aspettiamo alla prova dei fatti, non smetteremo di incalzarvi, lo faremo da forza di opposizione responsabile, che farà sempre il tifo per l'Italia anche dai banchi dell'opposizione. È con questo spirito che annuncio il voto di astensione di Azione-Italia Viva.

hanno partecipato, anche nella scorsa legislatura, all'impegno politico sul PNRR e tutti abbiamo condiviso, anche in momenti differenti o comunque con accenti diversi,

per dare addosso al Governo e alla maggioranza, accusando l'Esecutivo di incapacità, di caos e di perdita di finanziamenti. Tutto falso.

un approccio diverso, che deve guardare a due fattori in particolar modo: il realismo e la flessibilità. È quello che in questi mesi ha fatto il Governo. Questi due principale del Governo, con la possibilità oggi di rimodulare il PNRR e di renderlo quanto più attuale e attinente alla realtà di oggi, proprio per rilanciare l'azione attraverso una revisione

nelle settimane trascorse. Voglio cogliere un aspetto importante che forse dimentichiamo o trascuriamo. Il PNRR del nostro Paese è quantitativamente il più imponente e il più importante di tutta l'Europa. Immaginate

costruttivo con l'Europa proprio per chiedere condivisione e maggiore flessibilità, come riconosciuto anche dall'attuale commissario europeo Gentiloni, che di certo non ha la tessera di Forza Italia e che a sua volta afferma oggi la necessità di una maggiore flessibilità.

che queste sono risorse per investimenti e che ogni euro speso e convertito in investimenti genera un moltiplicatore che è ben diverso da quello della spesa improduttiva dell'assistenzialismo, forse tanto grato e tanto amato da qualche forza politica di opposizione. La nostra è una visione molto diversa rispetto a quella dell'opposizione, perché da sempre il nostro faro, il faro di Forza Italia e delle forze politiche di centrodestra, sono le politiche di investimento, per cui abbiamo oggi

figli. Siamo oggi fiduciosi e ottimisti sul raggiungimento di un accordo a livello europeo, sulla flessibilità e soprattutto sulla bontà

essere incapaci; invece io ritengo e noi riteniamo che sia un atteggiamento di grande responsabilità, di lungimiranza, di realismo e di credibilità che questo Governo e questa maggioranza hanno oggi nel Paese.

Non dobbiamo assolutamente drammatizzare, ma essere fiduciosi. Ce la stiamo mettendo tutta; ci sono progetti infrastrutturali molto importanti, che possono rivoluzionare e cambiare l'aspetto del nostro Paese, soprattutto cambiarlo in meglio, come tutti noi vogliamo e chiediamo.

Signora Presidente, ringrazio il Ministro per la sua presenza qui in Aula e in tutti i lavori della Commissione. È giusto dirlo: lei è stato sempre presente in Commissione e di questo la ringraziamo. Colleghi, siamo già alla votazione finale e quindi non vorrei perdermi nello scaricare o addebitare responsabilità a questo o a quell'altro Governo,

c'è una produzione così copiosa di norme, è chiaro che le soluzioni ancora non sono state individuate, per le difficoltà che si sono presentate. I dati sull'attuazione del PNRR li conosciamo tutti e li abbiamo letti tutti sui giornali; abbiamo letto pure la relazione della Corte dei conti. Il raggiungimento degli entro giugno 2026 e lo sblocco delle rate semestrali da parte dell'Europa (non mi riferisco solo a quella di oggi, che avverrà ad aprile, ma anche a quelle successive) sono tutti argomenti che agitano il sonno della maggioranza e lo capiamo, ma agitano pure tutti gli italiani e anche le opposizioni. Questo lo sappiamo, l'avete già detto, non è l'ultimo intervento normativo risolutore, ma non possiamo mica permetterci lunghi percorsi di riflessione per decidere la rimodulazione del PNRR, come molti ieri hanno detto in quest'Aula, tra i banchi della maggioranza. In Aula e in Commissione abbiamo sviscerato e snocciolato - anche i giornali lo hanno fatto - tutte le difficoltà che in questo momento si hanno per l'attuazione del PNRR, ma purtroppo abbiamo anche ascoltato frasi fatte,

poiché vengo dalla Sicilia: mannaggia, i soldi non li sapete spendere; allora, li prendiamo noi che siamo più bravi. Questa è una frase che si è ripetuta troppo spesso tra i banchi della maggioranza e mi ha un po' colpito. colpito. I problemi li abbiamo visti tutti, dall'inflazione ai bandi che faticano a vedere il traguardo, dal tema delle semplificazioni al problema delle liquidità, alle difficoltà dei Comuni. Però un punto fermo da cui partire, in quest'atto, per mettere

di coesione e il PNRR. L'accentramento e anche la riprogrammazione non riguardano però solo il PNRR, che ci sta tutto, ma soprattutto i fondi strutturali nazionali e anche regionali, senza considerare la politica di coesione, che prevede tre articoli all'interno dell'atto. Vorrei spiegare meglio questa mia affermazione, soprattutto quanto parlo dei fondi strutturali nazionali e regionali - lo specifico - perché forse nel decreto-legge

soprattutto all'emendamento presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia, che è stato riformulato dal Governo, con cui vengono riprogrammati i fondi strutturali nazionali, ma in cui si apre la porta anche a quelli regionali. L'intento non è chiaro o almeno io non l'ho capito. Lo spiego meglio ai colleghi, in modo tale che, se l'hanno capito, magari me ne possono dare contezza. L'emendamento in questione toglie i rimborsi oggi riconosciuti dall'Europa alle Regioni, a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, i cosiddetti progetti retrospettivi, ma rendicontati

riformulato dal Governo e approvato, si dice che questi rimborsi devono andare al fondo di rotazione per l'attuazione del cofinanziamento, per garantirne però poi, successivamente, la destinazione territoriale.

il senso di questa procedura? Sono stata alla Regione siciliana e credo che in tutta Italia le burocrazie non siano proprio così efficienti.

nel merito dei dettagli, si diventa vaghi e ambigui, soprattutto quando parliamo della dottrina dei vasi comunicanti. È vero, non abbiamo speso tutte le risorse della programmazione 2014-2020. È un dato di fatto e abbiamo troppi fondi a disposizione, europei e anche dei relativi cofinanziamenti. Però, cosa cosa accadrà in questa dottrina dei vasi comunicanti non è ancora chiaro, mentre dovrebbe esserlo, altrimenti ho il sospetto che non si tratti di nulla di buono per i territori più svantaggiati e, neanche a dirlo, per le Regioni del Sud. Questo perché i fondi strutturali regionali e la politica di coesione sono per il Sud. Si rivede la *governance* della politica di coesione con due o tre emendamenti, ma senza entrare nel merito dei dettagli, senza capire e comprendere bene un aspetto, il ruolo che avrà l'attività politica dei Governi regionali, la possibilità di indirizzo delle Regioni nell'individuare, all'interno dei piani di sviluppo e coesione, i progetti e le leve economiche che risolleveranno quei territori, con una partecipazione che avviene dal basso e non dall'alto. non dall'alto. Piani di sviluppo e coesione che, ad oggi, non sono pronti. Il piano di sviluppo e coesione 2021-2027 ancora non c'è e la colpa non è delle Regioni, ma del Ministero per il Sud.

Dove andranno a finire queste somme non spese? Nel piano di sviluppo e coesione 2021-2027? D'accordo, ma in forma aggiuntiva o a decurtazione di quanto già spetta alle Regioni? Il mio emendamento, che è stato ovviamente bocciato e ha avuto parere contrario, proponeva questo. Mi pare però che in Commissione questa tipologia di emendamento sia stata anche presentata non con la mia riformulazione, ma da altre forze politiche, tra cui la Lega, che trasformato in ordine del giorno per ben due volte, sia nel milleproroghe sia in quest'atto. Io però una risposta ancora non l'ho avuta, né in Commissione, né in Aula, e stiamo parlando di miliardi

come sa benissimo il vostro ministro Musumeci, che, fino a settembre 2022, insieme al Governo di destra-centro, ha governato la nostra Regione. Quindi, a lui vanno addebitate le responsabilità di non spesa, non ai cittadini siciliani! È vero, occorre riprogrammare e rimodulare il PNRR subito, ma la rimodulazione degli interventi dev'essere un'operazione chirurgica, ragionando progetto per progetto. Spostare i progetti che non potranno essere realizzati con il PNRR ad altri fondi di diversa natura comporterà il coinvolgimento di tutte le forze politiche nazionali e regionali, nonché delle parti sociali. Dunque, bisogna avere un atteggiamento non di accentramento politico, perché tutte le parti devono essere coinvolte, quando parliamo di programmi di sviluppo. Altrimenti, stiamo parlando di altro; altrimenti, c'è un approccio meramente ragionieristico dello spostamento delle risorse. In parole povere, occorre una visione di sistema Paese condivisa con tutte le forze politiche sociali, altro che accentramento. Ecco perché abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo permanente. Noi ci siamo, con un approccio, come lei ha detto ieri nella sua replica, serio e responsabile, ma dobbiamo vederci chiaro, dobbiamo vedere gli elementi, quindi sediamoci attorno a un tavolo e discutiamo di questa grande sfida, soprattutto perché con la dottrina dei vasi comunicanti ci saranno in campo più di 300 miliardi di euro e questo ovviamente accentua l'impegno di programmazione, di decisione e di realizzazione. L'approccio non può essere quindi ragionieristico: la *governance* la *governance* dev'essere più performante, affinché le risorse che vengono spostate siano allocate nel più breve tempo possibile, anziché in un tempo indeterminato.

che hanno natura addizionale anche rispetto alla destinazione dell'80 per cento della politica di coesione al Sud. Le possibilità di finanziamento che arrivano dall'Europa non sono più compatibili con i metodi della Cassa per il Mezzogiorno. L'accentramento della *governance* del PNRR - lo dice anche la relazione della Corte dei conti - complicherà il passaggio e quindi non ci sarà quest'accelerazione della spesa immediatamente, piuttosto ci sarà un rallentamento dell'azione amministrativa. Era proprio necessario in questo momento? Per noi il PNRR è una grande

Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, inizio con il chiarire che

l'attività parlamentare è stata premiata. Credo che la qualità dell'intervento parlamentare su decreti e, in generale, su testi di provenienza governativa dipenda dal numero degli emendamenti approvati. In questo caso, il numero degli emendamenti approvati (in senso *bipartisan*, perché sono stati approvati emendamenti della maggioranza e dell'opposizione) Dal punto di vista del lavoro in Commissione, non ho nulla da segnalare, se non aspetti positivi e un clima costruttivo e penso che questo sia veramente un grande miglioramento rispetto a quello che abbiamo visto nella scorsa legislatura, quando le contrapposizioni la maggioranza *pro tempore* e la minoranza *pro tempore* avevano un carattere totalmente ideologico. In questo caso, invece, mi sembra che il Parlamento sia valorizzato e invito tutti a proseguire così, perché è la maniera migliore.

che era messa in pericolo dall'ennesimo parco eolico regalato da Draghi alla Siemens, azienda tedesca senza nessuna

in questo caso sarà decisivo per riuscire a ottenere l'assegnazione del telescopio Einstein in Sardegna, con un enorme indotto per tutta l'isola.

Secondo voi, già tenuto presente qual è normalmente l'atteggiamento dell'Europa nei nostri confronti, una roba negoziata da Gualtieri potrebbe mai avere un senso economico-finanziario? Io direi di no, perché ovviamente è noto che non so per quale strano accidente della vita si era deciso di nominare come Ministro dell'economia qualcuno che l'economia non la sapeva,

perché si arriva a dire che il PNRR ha qualche problemino, cito un articolo di giornale dell'epoca (stiamo parlando del dicembre 2020) relativo all'incontro che il partito di Italia Viva, all'epoca parte della maggioranza, ebbe con il ministro Gualtieri. A una domanda dell'ex ministra Maria Elena Boschi sulla riforma della giustizia nella parte del PNRR relativa alle riforme di sistema, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri risponde candidamente che lui il piano non lo aveva letto.

di cosa parliamo. I famosi 200 miliardi, la pioggia di miliardi che è stata venduta, erano solo propaganda, erano solo una prima pagina del giornale «Il Fatto Quotidiano» per far vedere Conte con le banconote. Immagino che la ricordiate tutti, con le banconote che piovevano.

dei nostri risparmiatori, si trasferiscono nelle casse dell'Unione europea che ce li presta (quindi l'Unione europea ci presta i soldi dei nostri risparmiatori) con condizioni e con monitoraggi, vale a dire entrandoci in casa.

E poi vogliamo insegnare l'economia finanziaria nelle scuole? Forse dobbiamo iniziare a insegnare l'economia finanziaria a Gualtieri *(Applausi)*, almeno per capire di che diamine si parla; non dico a Conte, perché sarebbe una causa persa.

senza conoscere le condizioni e con tutte queste condizionalità, senza nessun tipo di dibattito parlamentare serio, è stato un azzardo epocale. Altro che le piccole cifre di cui discutiamo: praticamente il nostro Paese si è consegnato mani e piedi all'Unione europea, che controlla e guida quello che dovremmo fare con questi soldi, che poi alla fine sono nostri e non sappiamo a che prezzo li paghiamo, senza sapere come e perché. Tra parentesi

praticamente nessuna differenza sostanziale rispetto al nostro prezzo di finanziamento sui mercati. Non solo. Nessuno mi ha mai detto - e se per caso il Ministro lo sapesse, mi farebbe una cortesia a dirmelo - se questi prestiti sono privilegiati o meno, perché se per caso avessero le caratteristiche di credito privilegiato, pur avendo lo stesso prezzo del credito normale derivante all'emissione dei BTP, saremmo dei pazzi, saremmo dei pazzi, perché andremmo a prendere in prestito, a quelle condizioni, un credito che ha le caratteristiche di uno privilegiato.

di queste operazioni e per provare a fare più operazioni possibili nell'interesse dei nostri cittadini, ma l'importante è essere sempre sinceri con loro, altrimenti non potremo pretenderne il rispetto.

il lavoro del PNRR è certamente complesso; non invidiamo il compito del ministro Fitto, che ieri, nella sua replica - devo dire anche in maniera un po' piccata - ha criticato l'atteggiamento dell'opposizione, ma

sei mesi sono già un bel periodo per testare la direzione di marcia, il lavoro che volete fare e il percorso che legittimamente volete intraprendere. È evidente che a Bruxelles è scattato un *early warning*: quando ti danno 190 miliardi - magari rispondiamo anche al collega Borghi - evidentemente ci sono delle condizioni

in sede europea conta la credibilità, quindi se mantieni le promesse e se porti avanti le riforme promesse, legate agli obiettivi che dobbiamo cogliere ogni semestre in termini di investimenti e riforme. Ebbene, il rallentamento sulla riforma della competitività (leggi balneari) piuttosto che sulla giustizia ha fatto scattare e drizzare le antenne a Bruxelles. Non a caso, ci sono ritardi nell'assegnazione della cedola semestrale da 19 miliardi,

ha garantito quei margini di flessibilità che ci permettono di rimanere sulla linea di galleggiamento; però, quel tempo non lo dobbiamo sprecare. Abbiamo lavorato con senso di responsabilità al decreto-legge sul PNRR. E al ministro Fitto, ricordava il lavoro in Conferenza unificata, voglio dire che siamo tutti del mestiere, abbiamo avuto esperienze, lei stesso è stato Presidente di Regione e sa benissimo come funziona in quei consessi: si prova a costruire il consenso, ma non si è proprio tutti d'accordo. Si prova poi, con gli strumenti che ci sono - quelli classici dell'interlocuzione parlamentare - a proporre emendamenti che possano migliorare i provvedimenti. Ed è quello che abbiamo fatto con i colleghi della Commissione bilancio, con il capogruppo Daniele Manca, per trovare i meccanismi

che c'è un'esigenza di coordinamento, di accompagnamento del centro e di progetti complicati, anche per aggredire la criticità che lei giustamente ha ricordato ieri, relativa alla difficoltà di spendere da parte della nostra pubblica amministrazione, soprattutto in alcuni territori. Quei 18 emendamenti approvati, ministro Fitto, non sono una concessione alla minoranza per poi silenziarla in Aula e dire che non deve preoccuparsi di fare critiche al Governo. Noi rivendichiamo il nostro diritto-dovere di vigilanza e di controllo sulla vostra azione, come avete fatto voi quando eravate all'opposizione. Lo facciamo per questo, ma ancora di più perché, con orgoglio, siamo stati protagonisti di quella fase in cui

sosteneva il Governo Draghi, in cui abbiamo sostituito progetti che venivano finanziati proprio con il ricorso a debito delle aste dei BTP, che costavano decisamente molto di più degli eurobond. perché li abbiamo presi con la tripla A del *rating*; anche una persona che non ha fatto economia lo capisce, è molto semplice *(Applausi)* e il costo del debito è minore, altrimenti non si capisce perché andavamo a sostituire alcuni progetti che ci costavano molto di più con un debito che ci costerà molto di meno.

costruire i necessari equilibri con il Ministero dell'economia e delle finanze e non sarà facile; persone anche più strutturate in passato qualche problema l'hanno avuto; con Draghi ha funzionato, perché c'era un'integrazione fortissima fra i principali responsabili che lavoravano insieme da tempo. Ci sarà bisogno di una fase di rodaggio comprensibile e siamo preoccupati per i ritardi. attraverso il Presidente, mi rivolgo al ministro Fitto perché vorremmo capire quali sono i progetti che vengono cambiati. La seguiamo anche sul ragionamento relativo all'integrazione con i

capire con i sindaci di quei territori e delle comunità territoriali, che hanno costruito una *partnership* con le associazioni di categoria e con le forze sociali, per il rispetto che dobbiamo quali sono i progetti che cambierete. Entro il 30 aprile dovete dirlo e vorremmo saperlo, perlomeno rispetto ai 2,7 miliardi di Repower EU. Prima lo facciamo, meglio è, Ministro, perché, se vogliamo ricostruire e non accumulare ritardi, è bene che lo si faccia all'interno delle Aule parlamentari. Il presidente Conte e il presidente Draghi l'hanno fatto, sono venuti a riferire; poi scelga lei se vuole venire in Aula o nelle Commissioni competenti, bilancio e politiche comunitarie, ma ci si è confrontati sui progetti. Abbiamo discusso, abbiamo litigato anche all'interno delle forze di maggioranza se bisognava mettere più o meno soldi sulla sanità e noi siamo convinti che quella scelta sia stata corretta. Anche su Repower Eu, su quei 2,7 miliardi, possiamo aprire una discussione in Parlamento su dove metterli? Li mettiamo per contrastare la povertà energetica, li mettiamo per spingere sulle energie rinnovabili o per investire sulle comunità energetiche? Poco tempo fa, il presidente Prodi ha proposto l'idea, che è condivisa da molti, di provare a mettere in campo un progetto per coprire le aree industriali, commerciali e gli edifici pubblici col fotovoltaico, una politica industriale di sostegno alla filiera e un aiuto alle comunità locali, che possono risparmiare sulle bollette: aiutiamo famiglie e

femminile siamo davvero preoccupati per quella deroga prevista all'articolo 47, che era anche ragionevole. Sappiamo benissimo infatti che in alcuni settori, ad esempio nelle costruzioni, nell'edilizia e nell'ingegneria civile, è più difficile trovare figure femminili, ma noi abbiamo bisogno delle linee guida previste dall'articolo 47 del decreto n. 77 del 2021, e ce le avete tolte dall'ordine del giorno e dall'emendamento che avevamo proposto. Facciamolo, però, perché abbiamo bisogno di compensare il taglio, visto che in alcuni settori oggettivamente è difficile recuperare profili femminili già formati. Andiamo a compensare, definiamo misure premiali o sanzionatorie. Perché non lo facciamo? Aggiungo anche un'altra proposta:

ma siamo meno attenti all'impatto degli investimenti, attenzione che invece è presente nella cultura anglosassone. All'interno del Senato c'è un Ufficio di valutazione delle politiche pubbliche. Perché non ragionare insieme, non solo tra le forze di opposizione, visto che penso sia interesse anche delle forze di maggioranza, di una Commissione bicamerale con la logica dell'*investment review*? Andiamo a vedere se i progetti che mettiamo in campo incontrano le *milestone*, quindi le tappe intermedie e i *target*, ma soprattutto se vanno a cogliere l'obiettivo. Questo è uno strumento che aumenta la consapevolezza del legislatore e le scelte che dobbiamo fare noi e penso che sia utile anche al Governo. Pensateci, lo dico anche alle forze di maggioranza. Questo è l'approccio del Partito Democratico: critiche, mettiamo in evidenza quando siamo preoccupati dei ritardi, vogliamo conoscere quali sono i progetti che verranno cambiati, ma non verranno mai meno - perché abbiamo a cuore il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi del nostro Paese - le nostre le nostre proposte, perché questo lo dobbiamo al nostro Paese.

ai componenti della Commissione bilancio, in particolar modo ai due relatori, senatori Gelmetti e Testor, al presidente Calandrini e al Governo.

facendoci i complimenti per questo nuovo modello di comportamento istituzionale. Avevamo chiesto tutti insieme un protagonismo del Parlamento,

che deve informarsi un po' meglio, dev'essere più attento e deve trovare informatori un po' più attenti in 5a Commissione. Infatti, mentre lui diceva che i lavori erano impantanati, noi lavoravamo alacremente, ci confrontavamo con il Ministro

Abbiamo migliorato tantissimo il provvedimento, ascoltando tutti i componenti della Commissione, perché il Ministro ha avuto l'attenzione, la sensibilità e l'umiltà di ascoltare

PNRR e sui fondi che ci sono stati destinati quando il ministro Fitto, con estrema chiarezza, ha dichiarato che i criteri di assegnazione ai singoli Stati sono oggettivi. Non c'è stato un merito da parte di qualcuno, perché i criteri con i quali vengono distribuiti i soldi a ciascuno Stato

il modello dell'Agenzia, del non accentramento, come lo avete definito, perché pare che stiamo accentrando su Palazzo Chigi? Non riuscite a capire che nella misura in cui Palazzo Chigi chiede protagonismo,

ci mette la faccia, come tutto il Governo su questo provvedimento che avete disegnato e costruito voi nelle direttrici e noi, soltanto per senso di continuità istituzionale, lo stiamo difendendo

della responsabilità e del buon senso. Questo è quello che ha regalato il Governo Meloni a questa Nazione.

sulla storia del PNRR. È stata fatta oggi, con senso di responsabilità, per andare a verificare che le scelte sono state fatte da voi e i soldi sono arrivati per criteri oggettivi.

la controprova di tante situazioni e di tanti riscontri che ho sul territorio, ho la certezza che stiamo lavorando bene, assolutamente in discontinuità rispetto a chi ci ha preceduto. La terza rata arriverà, come ha detto Gentiloni, che ha compreso che deve cambiare atteggiamento nei confronti del Governo italiano.

lettere scarlatte al Governo affinché abbia meno potere contrattuale in Europa. Noi dobbiamo vestire tutti quanti la maglia azzurra. Lo so che questo colore non vi piace, ma dobbiamo vestire quella maglia *(Applausi)* che ci rende unici, migliori degli altri e più forti nella contrattualità.

date buoni consigli, quando non siete più in condizioni di dare il cattivo esempio grazie alle scelte degli italiani.

che stiamo vivendo; è quello che sta dimostrando il Governo Meloni ed è quello che sta dimostrando questa maggioranza, con senso di responsabilità. È questo atteggiamento che ci renderà più forti in Europa e nel mondo e che ci renderà credibili. È per questo che, con orgoglio e convinzione, caro Governo, cari Ministri e caro Sottosegretario, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia

ricordare in quest'Aula la strage di Primavalle, l'assassinio di Stefano e Virgilio Mattei. Lo facciamo perché domenica saranno cinquant'anni da quella notte del 16 aprile 1973, quando un gruppo di estremisti della sinistra extraparlamentare versò benzina sotto la porta dell'appartamento della famiglia Mattei, in via Bernardo da Bibbiena, e appiccò il fuoco. Quegli assassini non hanno mai pagato. Uno non c'è più, gli altri sono fuggiti all'estero da decenni. Domenica lo faremo anche in Campidoglio; stamattina, con Giampaolo, lo abbiamo fatto in una scuola (Giampaolo è il fratello, che con la sua associazione tiene viva la memoria dei fratelli e di quella strage). La strage di Primavalle colpì la famiglia di Mario Mattei, segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano, è stata uno dei crimini più orrendi di quegli anni. Erano gli anni delle stragi nere; c'era stata Piazza Fontana e, di lì a poco, ci sarebbero stati l'Italicus e la strage di Brescia. Anche il terrorismo rosso si stava affacciando sulla scena del crimine politico, con una scia di attentati e omicidi fino al 1978, l'assassinio di Aldo Moro e poi dell'operaio comunista Guido Rossa da parte delle Brigate Rosse. Erano gli anni dell'odio. In quel clima accadeva ogni giorno che, se un ragazzo aveva in tasca un giornale di destra, poteva venire aggredito; lo stesso per chi aveva in tasca "l'Unità" o un giornale con un titolo rosso, oppure indossava l'eskimo. Accadeva in tutta Italia. A Roma accadde anche a Primavalle: erano le ore 3,30, quella notte. C'è ancora la foto dei corpi carbonizzati di Stefano e Virgilio affacciati alla finestra a raccontarci cosa furono quegli anni. Quella foto - ha raccontato Giampaolo - per la famiglia non esiste, perché, ogni volta che veniva pubblicata, loro la tagliavano e lasciavano un buco sul giornale. Era troppo grande il dolore, troppo forte quell'orrore. Erano gli anni in cui un ragazzino di destra, Paolo Di Nella, di diciassette anni, venne ammazzato a sprangate perché attaccava manifesti. Pertini andò a trovarlo all'ospedale.

mi avvio a concludere questo mio breve intervento. Tante di quelle vittime, a Roma e in altre parti d'Italia, hanno visto intitolarsi strade o giardini. È un modo per contribuire a far sì che quella stagione dell'odio non ritorni. La memoria non può essere condivisa, ma dev'essere intera soprattutto, deve avere un denominatore comune. In politica ci dev'essere un avversario e anche aspra dev'essere la competizione, ma non devono esserci l'odio e la violenza. Questa è l'essenza della democrazia, che sta inscritta nella Costituzione e che ci apprestiamo a celebrare il prossimo 25 aprile.

e Carla Zappelli, la mamma di Valerio Verbano. Giampaolo è un "sacramento" di due metri, Carla Zappelli non c'è più, era una donna anziana e minuta. Ad un certo punto, vennero chiamati sul palco e si abbracciarono commossi: mondi diversi, che però erano uniti da un senso comune, per provare non a cicatrizzare ferite che non sono cicatrizzabili, ma a dire basta con quella stagione dell'odio. un gesto straordinario, per entrambi, anche con il rischio - poi accaduto - che i loro mondi di provenienza, quello dei fratelli di Giampaolo e dei figli di Carla Zappelli, non capissero fino in fondo quel gesto. È però

Grazie, senatore Verini. Sono questi i momenti in cui mi sento orgoglioso di presiedere questo Senato. La ringrazio veramente.

si ricolleghi anche alle parole con cui lei ha aperto questa legislatura, come ha detto poco fa il collega Verini, citando alcuni protagonisti di varie

sono impresse nella memoria della città, al punto che domenica ci saranno vari eventi, per ricordare questi cinquant'anni: uno sarà anche al Campidoglio, a cui io stesso parteciperò e ci saranno esponenti di varie aree politiche. Quindi è giusto ricordare, a cinquant'anni di distanza, quell'aprile del 1973 e il rogo di Primavalle, in cui la famiglia Mattei fu aggredita. Era un gruppo di Potere operaio che appiccò fuoco alla casa, con la benzina. Alcuni riuscirono a sfuggire a quell'attentato, ma Stefano e Virgilio morirono, due figli, uno un bambino e l'altro comunque giovanissimo. Io credo di essere l'unico, in quest'Aula, in questo momento, a poter dire che, a quindici anni, ho partecipato al funerale dei fratelli Mattei, nella chiesa di piazza Salerno.

A volte, la condivisione del ricordo non è stata facile nelle famiglie. Il senatore Verini parla di cose che conosce, perché ha svolto funzioni anche in Campidoglio. Sia familiari di destra sia di sinistra, che hanno partecipato a momenti condivisi, tuttora non trovano la comprensione intera della loro parte politica o delle loro famiglie. Succede. Io, che conosco queste famiglie, lo so per esperienza diretta. Io ritengo invece che si debba condividere la memoria. Presidente, molte cose si potrebbero dire, ma non è questa l'occasione. All'epoca, "Il Messaggero", che era il giornale più diffuso della capitale, come oggi, scrisse che vi era stata la faida interna dei missini. Vi fu addirittura un libro, che raccontò cose incredibili. Ci vollero anni per arrivare ai processi e anche il processo

questo era il clima dell'epoca. Un giornale importante pubblicava un libro e un'inchiesta che stravolgeva la realtà. Non c'era solo la violenza, quindi, ma a volte c'era anche la menzogna. Altri potrebbero citare diverse menzogne, ma non è il momento per fare l'elenco degli errori, bensì per ricordare questa storia. Lo faccio anch'io, con commozione, avendo conosciuto la famiglia Mattei, Giampaolo e tutti gli altri. E invito anche i familiari a condividere questi ricordi e queste memorie, perché questo serve per un processo vero di pacificazione nazionale.

in quella notte Stefano e Virgilio Mattei, rispettivamente di otto e ventidue anni, perirono nell'attentato incendiario provocato deliberatamente da figli di papà che giocavano ai rivoluzionari nelle file della sinistra extraparlamentare e che in quella notte di follia avevano deciso di dare fuoco alla povera abitazione di Mario Mattei, netturbino, con la sola colpa di essere il segretario della sezione del MSI Giarabub nel popolare quartiere di Primavalle. Mario Mattei riuscì miracolosamente a salvare se stesso, la moglie e gli altri figli, buttandosi giù dalla finestra di quella casa in cui dormivano in sette in tre vani, ma non Stefano e Virgilio, rimasti intrappolati dal fuoco. Una foto straziante ritrae i due corpi carbonizzati, con il più piccolo dei fratelli Mattei ancora abbracciato alle gambe del fratello più grande, in una disperata richiesta di aiuto. La follia di quegli anni racconta di vergognosi depistaggi, di tentativi della sinistra e della grande stampa di coprire e giustificare. Ignobile resterà la lettera di solidarietà di Franca Rame ad Achille Lollo, uno degli assassini. Altrettanto ignobile la campagna stampa di quei giorni, che tenterà di accreditare un'inesistente faida interna alla sezione di Primavalle: una ricostruzione vergognosa, smentita dalla sentenza della magistratura, che condannerà in maniera definitiva Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo

con gli assassini in libertà scappati in Nazioni compiacenti, che solo nel 2006 saranno rintracciati, ma che mai pagheranno davvero. Di quella orrenda strage si perse memoria fino al 2003, quando l'allora municipio XIX di Roma, che comprende il quartiere di Primavalle, decise di ricordare nel loro territorio i fratelli Mattei in quell'anniversario, intitolando loro un parco. Io ero consigliere comunale ricordo quella cerimonia con la svelatura della targa nel parco di via Battistini, seguita da una messa *in loco.* Alla toccante cerimonia parteciparono fra gli altri Federico Guidi e Marco Visconti, che vollero la targa, Teodoro Bontempo, Marco Clark, Domenico Franco, Marcello e Vilma Perina, Sergio Marchi, Marco Marsilio e tanti presidenti, assessori municipali dei municipi governati dal centrodestra, ma anche dal centrosinistra. Apprezzammo molto, senatore Verini, lo sforzo del sindaco Veltroni di porre un ricordo condiviso. Le violenze in quei giorni fecero cadere ragazzi di destra, fecero cadere ragazzi di sinistra. Qualche giorno dopo la cerimonia, quella targa fu sbrecciata da mani vigliacche, ma è ancora lì, come ancora lì è il parco Stefano e Virgilio Mattei, nella loro Primavalle. Da quell'anno, ogni anno, una cerimonia vuole ricordare quella strage. La mattina di domenica 16 aprile alle ore 10 le istituzioni nazionali, regionali, comunali e municipali ricorderanno Stefano e Virgilio Mattei in via Bibbiena. Una cerimonia, com'è stato appena detto, sarà celebrata in Campidoglio, a perenne monito, per ricordare l'odio criminale comunista, la vergognosa impunità e latitanza coperta degli assassini, la necessità di perseguire una giustizia ancora negata dalla latitanza dorata dei colpevoli e il sacrificio di Stefano e Virgilio Mattei, martiri di Primavalle caduti per l'Italia, affinché mai più una violenza così cieca possa bagnare di sangue la nostra Italia.

insieme a Iaio Iannucci, fanno sperare in quello che non è annullamento dei ricordi della storia, ma un modo diverso di ricordare, di affrontare e di condividere il senso di civiltà che deve accomunare tutte le parti politiche. Grazie veramente per oggi.

Grazie